la seduta era già stata tolta. Capisco che non c'era l'accordo delle componenti politiche, ma credo che un minimo di forme debba essere

anche a nome dei senatori che ho incontrato uscendo e che non sono riusciti a votare

Invito i senatori Segretari ad effettuare un rigoroso controllo.

si dà mandato al Ministero dello sviluppo economico per la definizione di indirizzi, in modo che possano essere affrontati quei temi che vanno precisati. La pregherei pertanto di tener conto di questa precisazione,

Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto anche per insistere nei confronti della relatrice rispetto al parere contrario espresso nei confronti di questo emendamento

con l'adozione di uno strumento come quello qui previsto. Mi riferisco alla creazione di un sistema che diviene una sorta di banca dati dei clienti finali

una questione così diffusa e delicata quale quella che fa capo agli elementi di garanzia del trattamento dei dati personali di così tanti utenti, che sono appunto gli utenti finali,

Presidente, sui subemendamenti relativi all'emendamento 1.0.7 vorrei richiamare l'attenzione della relatrice,

a Commissione serve semplicemente a celare una bastonata alle autorità indipendenti, imponendo loro non solo delle finalità generali, ma anche come devono conseguirle,

modificare la dizione «che può notificare» con quella, più appropriata, «che deve notificare». Avanziamo tale proposta per rendere certo il procedimento della Conferenza dei servizi, perché talvolta accade che, attraverso l'intento di velocizzare, le questioni possano risultare complicate, in quanto l'incertezza del procedimento apre lo spazio ad apprezzamenti di natura discrezionale che possono essere eccepiti dinanzi alle autorità competenti. Per questo motivo, dal momento che i Comuni entrano a pieno titolo nelle decisioni che devono essere assunte e che la stessa norma prevede la partecipazione diretta dei Comuni, la notifica deve costituire non un'opzione di natura procedimentale ma rappresentare una certezza. Per questo motivo, ci permettiamo di insistere perché il subemendamento venga preso in seria considerazione in modo da rendere certi i procedimenti e eliminare contenziosi e perdite di tempo.

la competenza delle questioni in oggetto. Il rischio che si è verificato - ne abbiamo già discusso in Commissione - è che un procedimento autorizzativo, detenuto esclusivamente per legge, così come adesso dirò, dal Ministero, possa essere paralizzato da un singolo Comune che è oggetto semplicemente di attraversamento della rete. Sapete che abbiamo un obbligo di sicurezza nazionale sulla trasmissione: questa proposta emendativa riporta appunto in capo al Ministero la possibilità di acquisire il parere degli enti locali. Voglio anche ricordare che il decreto-legge n. 239 del 2003,

con la legge n. 99 del 2009 abbiamo introdotto proprio qui in Senato la possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio attività per la realizzazione di varianti senza impatto localizzativo degli elettrodotti.

l'articolo 3 presenta una delicatezza che credo non sfugga a lei, né all'intera

sono precisamente descritte in quella legge. In quella circostanza disapprovammo quella decisione, perché a nostro parere l'Agenzia, per come veniva costituita, non avrebbe avuto quella autorevolezza che pure la questione avrebbe meritato. A questo scopo presentammo numerosi emendamenti perché l'Agenzia potesse costituire un fattore di garanzia per il Paese, indipendentemente dalle valutazioni di ciascuno circa l'opportunità di tornare al nucleare piuttosto che continuare con altre fonti energetiche. L'Agenzia avrebbe dovuto rappresentare un fattore di garanzia per il Paese. La maggioranza ritenne di non accettare le nostre proposte, i nostri emendamenti, e fu varata quella norma che oggi si decide di modificare riducendo ancora l'autonomia della stessa Agenzia. Si ritiene di modificare quella norma non essendo, peraltro, intervenuti fatti nuovi da allora ad oggi, in questi quattro mesi, e creando una situazione di oggettivo imbarazzo, perché il Parlamento ha la titolarità nell'esercitare una funzione di indirizzo, di controllo, nell'esercitare anche una attività tesa ad esprimere un giudizio sull'attività di questi organismi. Ed è facile immaginare quale situazione imbarazzante si determinerebbe nel momento in cui il Parlamento fosse chiamato a pronunciarsi su atti che vedono la piena titolarità e responsabilità di un proprio membro, e con quale imbarazzo la maggioranza o l'opposizione si troverebbero a valutare le questioni di merito; imbarazzo nel senso di

per esercitare l'alta funzione di governo di un'Agenzia che non è organo di indirizzo politico ma tecnico, che deve appunto garantire quella terzietà che l'apprezzamento di natura tecnico-scientifica può garantire, pur nel quadro di opinioni diverse e plurali che si possono mettere in campo. Segnaliamo quindi con forza questo problema e vorremmo che al nostro Paese venisse risparmiato questo ulteriore scivolone, che certo non farebbe crescere il nostro posizionamento nella comparazione con i Paesi che purtroppo ci sopravanzano, pur avendo alle spalle minore e meno gloriosa tradizione di civismo, democrazia e anche di maturità nell'esercizio delle funzioni democratiche e nella garanzia dei diritti di tutti attraverso le posizioni plurali ed autorevoli che le autorità indipendenti normalmente garantiscono.

tecnologie che consentano l'integrale cattura e sequestro del biossido di carbonio, l'anidride carbonica. L'Europa ci chiede di fare in tutto il continente dodici di questi impianti; uno di essi può trovare una localizzazione ideale in Sardegna, in cui sono presenti le uniche miniere di carbone del nostro Paese. Purtroppo, però, da circa un anno la norma che fu inserita nella legge n. 99 non ha trovato alcun tipo di attuazione. Gli emendamenti che vi chiediamo di approvare Governo in condizione di negoziare al meglio con l'Unione europea il sistema di realizzazione

del 2009, chiedo di prendere atto della cancellazione della disposizione riguardante la copertura finanziaria perché, come giustamente ci ha fatto osservare la Commissioni bilancio, non ce n'è bisogno.

che porterà il gas metano dall'Algeria all'Italia e poi in Europa, passando per la Sardegna, si preveda un meccanismo di compensazione per i costi extra legati all'utilizzazione dei derivati del petrolio.

ai giornali italiani: Parco marino nel golfo degli Angeli davanti alla spiaggia del Poetto; l'azienda fa richiesta al Ministero delle infrastrutture. Manifestazioni di piazza, *caos* incredibile. Dice l'amministratore con tono stizzoso: «Non vi è stata alcuna resistenza al nostro progetto da parte della Regione per il semplice motivo che non abbiamo avuto rapporti con loro.

Egli non negherebbe di aver ricevuto pressioni di tipo politico, ma avrebbe spiegato ai magistrati di non aver mai ceduto; avrebbe sempre cercato di rinviare l'adozione di atti che gli venivano chiesti, pur senza rompere con i referenti romani del partito, tanto che l'adozione delle delibere antieolico nel marzo 2010 sarebbe frutto di un lavoro iniziato nell'ottobre 2009 a causa della legge che noi vogliamo modificare.

per dare risposte alle loro popolazioni e non riconoscere che abbiamo fatto un errore ad immaginare che questo tipo di impianti possa venir autorizzato senza alcuna interlocuzione da parte delle Regioni italiane? Lo dico alla senatrice Vicari: siamo anche disponibili, tanto per iniziare la riflessione, a modificare l'emendamento, riportando una competenza delle Regioni, a partire da quelle a Statuto speciale, ma bisogna ricominciare ad essere realisti nell'immaginare la funzione dello Stato e di tutte le altre autonomie locali su queste vicende.

non siamo ancora in grado di intervenire, perché il nostro Paese non ha costituito le Autorità di bacino distrettuali: siamo ancora fermi alle Autorità di bacino *ante* concordato con il Ministero dell'ambiente, si chiede semplicemente di delegare, senza aumento di spesa per lo Stato, le attuali e già costituite Autorità di bacino ai ruoli che invece saranno successivamente destinati

sanzioni a livello comunitario. Questo è il contenuto dell'emendamento, che ci tenevo ad illustrare perché francamente non riesco a comprendere per quale motivo si paventi il rischio di un aumento di costi per le casse dello Stato, e neppure comprendo per quale motivo

dell'incompatibilità consentendo anche ai parlamentari di rimanere in carica anche dopo aver assunto determinati tipi di posizione - una situazione grave di per sé, ma ancora più grave in un contesto in cui i parlamentari non sono necessariamente espressione del territorio o magari di riconosciute capacità o onori acquisiti sul campo della politica, perché sono meramente espressione dei vertici dei partiti - riteniamo che vi debba essere almeno obbligatorietà di determinati tipi di passaggi parlamentari nel massimo della pubblicità. Dunque, comunque sia, pur riconoscendo

presentatori di ritirarlo e di trasformarlo in ordine del giorno.

presentata dalla senatrice Bonino, sono anche inaccettabili nel merito. Azzerare le incompatibilità previste per il presidente ed i membri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, stabilite tra l'altro dalla legge istitutiva varata pochi mesi fa dal Governo e dalla maggioranza, ed azzerare per il presidente persino l'incompatibilità con incarichi elettivi, significa contraddire le funzioni assegnate a questo organismo dalla maggioranza e dal Governo. Questo è un organismo che dovrebbe essere il principale garante di un'informazione corretta e trasparente ai cittadini su tutte le materie connesse alle tecnologie nucleari, dal funzionamento di eventuali nuove centrali allo smaltimento delle scorie. È nota la contrarietà del PD al programma nucleare varato da questo Governo, ma in questa occasione faccio finta di non pensarla così e di essere anche io un fautore convinto del ritorno al nucleare. tutto si può dire del nucleare tranne che non sia un'opzione largamente controversa nell'opinione pubblica. Allora, il principale compito dell'Agenzia dovrebbe essere di rassicurare i cittadini, proponendosi come garante credibile e autorevole della sicurezza. La prima preoccupazione di chi sceglie i vertici di questo organismo dovrebbe essere di indicare figure indipendenti che rispondano soltanto a questo ruolo e non anche ad altri ambiti di rappresentanza, a cominciare da quelli propriamente

Governo - un parlamentare notoriamente favorevole al nucleare (come immagino) sarebbe la negazione di una sua funzione effettivamente terza rispetto al Governo e alle imprese che saranno coinvolte nel *business* nucleare. Da antinuclearista convinto (secondo qualcuno anche ideologico), sarei tentato di augurarmi che commettiate questo errore, perché per me sarebbe molto più facile sostenere che questo nucleare è una bufala, è una scelta - come avrebbe detto Ennio Flaiano - grave, ma non seria. Ma siccome più ancora che al no al ritorno al nucleare, sono affezionato alla dignità delle istituzioni, vedo in questa proposta un altro passo verso la sistematica negazione dei principi della separazione dei poteri e della necessaria terzietà degli organismi pubblici di garanzia. Per questo invito tutti i colleghi a votare a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3.

non solo il ruolo dell'Agenzia merita qualcuno che ci si dedichi a tempo pieno, ma vorrei aggiungere, molto sommessamente, che anche la funzione di parlamentare merita qualcuno che ci si dedichi a tempo pieno.

incompatibilità, almeno andrebbe consentita la possibilità di far conoscere, con sedute pubbliche, da convocarsi prima delle decisioni, ciò che si dovrà poi subire senza avere alcun modo di opporvisi, relativamente alle decisioni che verranno assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quindi, si chiede semplicemente, al comma 8, al quarto periodo, di sostituire le parole «possono procedere» con «procedono» e di inserire dopo la parola «audizioni» la seguente: «pubblica».

Presidente, siamo perplessi rispetto alla pronuncia della Commissione bilancio che ha inteso

alla luce delle seguenti, rapidissime, motivazioni. L'attuale disciplina fiscale in materia di accise sui consumi di energia per usi non domestici penalizza fortemente i consumi inferiori a 200.000 chilowattora al mese. Il gettito complessivo per l'erario è pari a circa un miliardo di euro all'anno interamente a carico delle piccole e medie imprese comprese in tale scaglione di consumi. La nostra proposta intendeva redistribuire il carico fiscale tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese energivore, eliminando così un effetto distorsivo della fiscalità energetica sulla concorrenza tra sistemi di imprese. Un'operazione dall'impatto finanziario neutro per il bilancio pubblico, perché ci sarebbe stata, appunto, una compensazione tra sistemi imprenditoriali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

a valutare l'opportunità di assumere queste determinazioni in uno dei prossimi provvedimenti. Ciò, al fine di pervenire ad un riequilibrio dell'imposizione fiscale in campo energetico tra le piccole e medie imprese, oggi fortemente penalizzate, e gli altri sistemi di impresa.

Sanna che a settembre sarà depositato in Parlamento il disegno di legge annuale sulla concorrenza, nel quale sarà dato ampio spazio al settore energetico,

un interesse particolare per quanto riguarda il tema dell'energia da parte della criminalità organizzata. In Sicilia, ma anche in molte altre parti del territorio, ci sono già pale eoliche che non sono collegate; ci sono pale eoliche che potrebbero produrre più energia di quella di cui la Sicilia ha bisogno: rischiamo di far decollare la Sicilia con le sole pale eoliche. credo sia importante ribadire che l'energia è un bene essenziale per la vita dei cittadini, per le imprese e per i servizi, ha un suo valore strategico ed anche politico, è un elemento indispensabile per la qualità della vita. Spesso, lo sviluppo del territorio è dipeso dalle diverse scelte operate dai Governi nazionali e locali: la gestione privata dell'energia ha spesso privilegiato territori, aree, imprese, attuando gestioni oggettivamente né democratiche, né trasparenti. In questo testo, non si evidenziano risorse pubbliche da investire. C'è un rischio che bisogna evitare, abbiamo presentato emendamenti (anche l'emendamento 1.11), allo scopo di impedire discriminazioni territoriali e di affermare il valore della democrazia economica privilegiando il ruolo pubblico per mantenere

abbiamo sentito invece qui il sottosegretario Jachino.

che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno segnalato ripetute volte al nostro Paese e che sicuramente ha un impatto non trascurabile sulla libertà economica e sull'animazione dei mercati dell'energia, e in modo particolare del gas. Con questo emendamento riproponiamo, quindi, la separazione proprietaria nella gestione del trasporto e dello stoccaggio del gas rispetto agli operatori del settore. Per questo motivo, poniamo ancora una volta la questione, nella speranza che questa maggioranza voglia compiere un atto liberale a favore della nostra economia.

Rispondo solo con una frase al senatore Sanna, che prima ha detto che in Sardegna c'è un presidente che è sotto pressione. Voglio solo dire che nei quattro anni e mezzo della Giunta Soru si è subita un'azione forte nei confronti della Giunta regionale, sino a creare delle condizioni tali per cui, grazie del nostro Paese controllava totalmente l'energia alternativa in Sardegna; mentre posso dire, per quanto riguarda invece questa stagione, che vi sono iniziative per controllare che non ci sia un'avanzata degli speculatori in Sardegna, che hanno visto protagonisti senatori come me, come il senatore Quagliariello, come il senatore Massidda e come tanti deputati della Repubblica italiana del centrodestra, che si sono impegnati affinché in Sardegna ci sia un monitoraggio costante, ad evitare uno sbarco degli speculatori. Grazie a noi si è evitato anche questo.

di poter apporre la propria firma ad un emendamento del quale anch'io sono firmatario. Il collega Sanna ed io accettiamo questa richiesta, con la necessità impellente, però, di chiarire che non accettiamo le motivazioni che il collega Sanciu propone. Senza che io abbia bisogno di rendermi interprete delle affermazioni testé rese dal senatore Sanna, credo che vada comunque ribadito, signor Presidente, che ciò che il collega ha voluto dire, e che io in questo momento ribadisco, non è né una forzatura della realtà, né un'interpretazione soggettiva, tanto meno la ricerca di un elemento di

visto che il collega Sanciu ha voluto farvi cenno, stiamo vivendo una situazione istituzionale assolutamente drammatica. Abbiamo un Presidente della Regione reo confesso di "babbeismo". il Presidente della Regione sarda, di nome Cappellacci, si è definito babbeo: ha detto ai magistrati e ai giornalisti che lo hanno intervistato di essere stato un babbeo nel ricevere ed accettare regolarmente gli inviti di un signore che si chiama Flavio Carboni. Allora, collega Sanciu, se si ha il buon gusto

lei, per nascondere le vergogne di Cappellacci, pretende di offrire, in maniera fraudolenta, un'immagine dell'ex presidente Soru diversa da quella che è stata, introduce elementi di scorrettezza politica.

Presidente, non è questa la sede per siffatte gravi scorrettezze: attaccare delle persone che non sono in condizioni di difendersi perché non partecipano a quest'Assemblea.

Presidente, io intendo riconfermare che questa è una copertura che fu posta in via assolutamente prudenziale per evitare ragionamenti come quelli che si stanno oggi proponendo. Si tratta di una mera proroga di termini e non vi è nessun onere a carico dello Stato.

da parte del Governo si comunicò come urgente ed indifferibile la necessità di modificare il regime degli incentivi. A questo riguardo, numerosi programmi che peraltro avrebbero potuto utilizzare risorse comunitarie sono stati rallentati, se non addirittura paralizzati, con evidenti ricadute negative per le aziende e con il rischio di perdere le risorse comunitarie. Per questa ragione noi riteniamo che esistano tutte le condizioni perché il Ministero dello sviluppo economico, privo di titolarità in apparenza,

slittare ancora di ulteriori diciotto mesi il varo della riforma degli incentivi significa paralizzare e frenare la pur timida crescita che in questi ultimi tempi si evidenzia, che viene particolarmente enfatizzata e che noi vorremmo fosse sostenuta

avremmo difficoltà a votare a favore di questo provvedimento. Per quanto riguarda l'articolo 3

Cito solo l'emendamento 1.0.5, che è esemplare di come si legifera sugli argomenti.

«che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti». Non si vieta a chi non può fare gli impianti di avere l'autorizzazione, ma si chiedono congrue garanzie finanziarie, quelle che quotidianamente qualsiasi banca fornisce a chi interviene nel settore, e siffatti procedimenti sono consentiti non solo ai soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione, ma persino ai subentranti.

Si prevedono altri sei mesi per completare le procedure che dovrebbero consentire alle regionali di Sviluppo Italia - per capirci - di passare dallo Stato alle Regioni.

e parenti di parlamentari, consiglieri regionali, segretari di partito, e tutti sono coinvolti. Con grande onestà voglio dirvi che con sofferenza non potrei votare a favore di questo emendamento in nessun caso. Lo trovo oggettivamente, ancor di più in questo periodo,

ai motivi per cui siamo contrari. Il primo riguarda il costume, ormai invalso, di tornare su provvedimenti adottati in fretta, male, bocciati dalla Consulta su cui si interviene in seconda battuta cercando di pasticciare il più possibile ciò che era già pasticciato. Il secondo motivo riguarda il rifiuto del criterio della straordinarietà. Alcuni emendamenti da noi presentati riguardavano, appunto, l'idea che in nome della straordinarietà si compiono scelte sbagliate, frettolose e su cui si deve ritornare.

veniamo al quarto motivo, che è un corollario del terzo), in caso di mancato accordo tra Governo e Regioni, si stabilisce la supremazia di una delibera del Consiglio dei ministri che

A tal proposito ricordo che, in disaccordo con questo punto di vista, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato un ordine del giorno a prima firma Bugnano con cui si invita il Governo a fare tutto il possibile per evitare di lasciare margini di dissidio significativi tra Regioni e Stato in modo da poter poi rinunciare anche a questa potestà sovraimposta. Il quinto motivo è la caratura interna della pratica emendativa, al cui interno sono stati inseriti numerosi elementi che riguardano temi di natura energetico-ambientale che sono, in realtà, più ambientali che energetici: quindi, in un certo senso, in contrasto con la sostanza e il titolo del provvedimento. Come sesto punto,

Il settimo punto riguarda l'oggetto misterioso dell'emendamento x1.0.1, che per noi è del tutto e massicciamente improponibile,

contenute delle disposizioni di carattere ordinamentale incompatibili con un provvedimento d'urgenza. Senza fare troppi giochi di parole, la materia di questa incompatibilità è proprio

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, mi preme evidenziare che il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2009 sui commissari straordinari. Ancora una volta il Governo aveva ritenuto che l'unica via percorribile per dotare l'Italia di infrastrutture energetiche efficienti fosse la designazione di alcuni commissari straordinari. La necessità di procedere alla loro nomina era infatti emersa lo scorso anno ed aveva come obiettivo la realizzazione di interventi urgenti nel campo delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle reti di trasmissione dell'energia. La Corte costituzionale, però, ha ritenuto illegittime le richiamate norme, giudicandole in contrasto con le competenze delle Regioni in materia di energia e giungendo all'ennesima fase di stallo istituzionale in campo energetico. Apprezziamo comunque l'idea di fondo del Governo di ampliare il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per produzione, distribuzione e trasmissione dell'energia, ma denunciamo l'eccessivo ricorso a ruoli di carattere straordinario ed emergenziale anche quando sono superflui. Il nostro Paese sta conoscendo anni di continue emergenze senza che venga mai presentato un piano pluriennale di interventi concertato con gli enti locali, ma, allo stesso tempo, rigido ed efficace. È nostro dovere, quindi, verificare tutti i requisiti di straordinarietà ed i relativi effetti giuridici, proprio perché il provvedimento è emanato per ovviare ad un giudizio di costituzionalità. Concordiamo però con lo sforzo del Governo orientato a migliorare il livello infrastrutturale energetico del Paese, ma richiediamo che la parola chiave di tutto sia la concertazione con gli enti locali, con tempi certi e risultati chiari. Altro motivo di preoccupazione è la mancanza di una guida unica del Ministero dello sviluppo economico, che versa ormai da mesi in un limbo interinale non degno di un Paese di un Paese efficiente. D'altra parte, dal momento che è nostra abitudine evidenziare anche le iniziative positive del Governo, vorrei sottolineare che il nostro Gruppo apprezza anche che si fissi al 31 dicembre 2010 un termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle Regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Concludo domandandomi quale sia la motivazione che ha portato all'ampliamento dei poteri di controllo e di vigilanza del Ministero per la semplificazione normativa nel processo di nomina e revisione dei commissari straordinari, auspicando che non sia una lottizzazione mascherata interna alla maggioranza. A nostro giudizio, è evidente che ci sono ancora troppi nodi da sciogliere e troppa poca chiarezza, non tanto sugli obiettivi che il Governo si è prefissato, quanto sul modo in cui conta di raggiungerli. Per queste motivazioni, il nostro voto sarà contrario.

intervengo per annunciare il voto contrario del Partito Democratico, come era facile evincere anche dagli interventi che abbiamo pronunciato sui singoli emendamenti. Le ragioni sono evidenti. L'articolo 1 disattende il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale e, a nostro parere, si espone a possibili ulteriori contenziosi perché non si precisa esattamente in quali circostanze possano essere invocate le ragioni dell'indifferibilità e dell'urgenza e diventa anche difficile qualificare come indifferibili ed urgenti interventi che appartengono all'ordinaria attività nella gestione e nella garanzia di servizi energetici per il nostro Paese.

che sicuramente verranno espressi dagli autorevoli colleghi nel caso in cui il Governo intendesse avvalersi della deroga che si rende praticabile di una decisione grave, proprio a fronte di una questione che avrebbe meritato invece il massimo della terzietà, e soprattutto chi ha sposato le ragioni del nucleare avrebbe dovuto offrire al Paese quegli elementi di garanzia che con tale norma vengono meno. Per tale motivo, siamo fortemente preoccupati per la tutela degli interessi generali del nostro Paese.

Grazie all'attenzione e all'impegno della relatrice, senatrice Vicari (che vogliamo ringraziare), numerose questioni importanti sono state inserite, e su di esse abbiamo espresso

non è qualificabile soltanto in termini di assenza fisica, ma è risultata evidente soprattutto per l'assenza di indirizzo politico.

norme stabili per offrire certezze al sistema produttivo, ad un mercato che deve poter dispiegare il massimo dei benefici per le imprese e per i cittadini, e agli investitori. Ancora una volta si perde un'occasione importante per offrire un contributo per il rilancio dell'economia nel nostro Paese e per contrastare la grave situazione di crisi; ancora una volta esprimiamo il nostro rammarico, pur avendo manifestato nei lavori in Commissione ed in Aula il massimo impegno per contribuire a migliorare un testo che avrebbe richiesto ben altra attenzione da parte del Governo e della maggioranza.

Sono vicende che sono state segnalate nell'interrogazione presentata in data 23 marzo 2010, sollecitata nel maggio 2010 e risollecitata oggi, anche per gli aspetti di carattere penale che coinvolgono la sicurezza dei lavoratori, i posti di lavoro, la sicurezza degli impianti e della popolazione.

che esiste la tessera del tifoso. Non esiste nessuna tessera del tifoso, né esiste una norma di legge, ma soltanto delle ordinanze che in qualche modo impongono un certo tipo di comportamento. Esiste sì un disegno di legge del senatore Benedetti Valentini in 1a Commissione, occorrerebbe portarne a termine l'esame di quel disegno di legge prima di passare alle dichiarazioni, affinché non siano confusionarie come quelle che invece occupano i giornali. **Sulla

Ho voluto fare questa comunicazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché da mesi sollecitiamo un intervento significativo che riguardi l'amministrazione penitenziaria, la polizia